Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta del 3 novembre 2009, ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide: per la Regione Sicilia: Benedetto Adragna, Bruno Alicata, Antonio Battaglia, Enzo Bianco, Sebastiano Burgaretta Aparo, Roberto Centaro, Vladimiro Crisafulli, Salvatore Cuffaro, Antonio D'Alì, Gianpiero D'Alia, Mario Ferrara, Giuseppe Firrarello, Salvo Fleres, Vincenzo Galioto, Costantino Garraffa,

per la Regione Veneto: Maria Elisabetta Alberti Casellati, Anna Cinzia Bonfrisco, Federico Bricolo, Luciano Cagnin, Felice Casson, Maurizio Castro, Franca Donaggio, Alberto Filippi, Maurizio Fistarol, Paolo Franco, Mariapia Garavaglia, Paolo Giaretta, Elio Lannutti, Pietro Longo, Enrico Morando, Paolo Nerozzi, Luigi Ramponi, Maurizio Sacconi, Maurizio Saia, Paolo Scarpa Bonazza Buora, Piergiorgio Stiffoni, Marco Stradiotto, Gianvittore Vaccari, Gianpaolo Vallardi; per la Regione Lazio: Laura Allegrini, Andrea Augello, Paolo Barelli, Giuseppe Ciarrapico, Angelo Maria

Marino, Riccardo Milana, Stefano Pedica, Marcello Pera, Raffaele Ranucci, Oreste Tofani, Vincenzo Maria Vita e Luigi Zanda; per la Regione Puglia: Francesco Maria Amoruso, Antonio Azzollini, Giuseppe Caforio, Gianrico Gianrico Carofiglio, Rosario Giorgio Costa, Luigi D'Ambrosio Lettieri, Cosimo Gallo, Luigi Grillo, Nicola Latorre, Simonetta Licastro Scardino, Alberto Maritati, Salvatore Mazzaracchio, Colomba Mongiello, Carmelo Morra, Pasquale Nessa, Adriana Poli Bortone, Donatella Poretti, Giovanni Procacci, Michele Saccomanno, Alberto Tedesco e Salvatore Tomaselli. Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate tali elezioni. Informo, inoltre, che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta del 3 novembre 2009, ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide: per la Regione Piemonte: Tomaso Zanoletti; per la Regione Friuli-Venezia Giulia: Vanni Lenna. Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate tali elezioni.

la complessità del decreto-legge in esame può indurre ad abusare, una volta di più, della lingua di Cicerone, quale disinvoltamente si attinge per etichettare quei provvedimenti caratterizzati dal contenere di tutto un po', senza soverchie pretese di organicità e coerenza, come è stato evidenziato dagli interventi che mi hanno preceduto e dalla relazione sulle questioni pregiudiziali di questa mattina. Ad onor del vero, in questo caso non credo che la definizione di *omnibus* sia la più consona poiché il fattore preponderante e, in qualche modo, unificante del provvedimento, esiste, ed è offerto dalla premura obbligata di adeguare il nostro ordinamento a quanto promulgato in sede europea, nonché di sanare trasgressioni e inadempienze correlate a procedure pendenti di infrazione comunitaria. Azioni sanzionatorie, queste ultime, a volte innescate da questioni magari non trascendentali (e potremmo farcene un'idea dalla materia di di una delle ultimissime procedure di infrazione giunta a carico dello Stato italiano, che risponde al titolo: «Ostacoli all'uso dei bagni mobili chimici), dei bagni mobili chimici), che tuttavia danno origine a contenziosi la cui onerosità rende altamente consigliabile una solerte soluzione. E tale considerazione, sia detto per inciso e senza intento polemico, dovrebbe forse sollecitare una ragionevole continenza nella produzione di emendamenti. Vorrei ricordare che poco più di un mese fa, il numero totale delle procedure di infrazione a carico dell'Italia si attestava a 155, di cui 125 concernenti casi di violazione del diritto comunitario mentre le restanti 30 attinenti a mancata trasposizione di direttive nell'ordinamento italiano. Ho presente che ai tempi del Governo Prodi, appena tre anni fa, l'Italia svettava nella classifica europea delle infrazioni comunitarie con 274 procedure aperte, di cui ben 80 soltanto in materia ambientale: è avvenuto proprio con un Esecutivo di sinistra che sfoggiava un "verde" nel ruolo di Ministro dell'ambiente. Violazioni ed inosservanze in ambito ecologico, d'altro canto, conservano tuttora il primato numerico, sebbene ampiamente ridimensionato, e certo non mancano di caratterizzare, dal punto di vista dell'intervento risolutore, l'Atto Senato n. 1784 che veicola il decreto-legge 25 La materia ambientale, così, ricorre in diversi articoli, dal trattamento dei mezzi di locomozione fuori uso alla promozione delle innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente e all'abbattimento delle emissioni, dalla riduzione dell'uso delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche al loro smaltimento ecologico, sino alle nuove disposizioni tributarie relative alle imposte di consumo sugli oli lubrificanti rigenerati. Credo, pertanto, che le accuse di eterogeneità vadano ridimensionate rapportandole all'intrinseca natura "riparatoria" del provvedimento e, in ogni caso, debbano considerarsi la sussistenza di indiscutibili colonne portanti, quali - appunto - la vocazione ecologista che ne caratterizza in maniera preponderante la finalità. Il lavoro dei senatori ha poi consentito di ampliare la portata del decreto-legge, spaziando anche su questioni connesse connesse alla già manifestata connotazione ambientale, quale l'adeguamento della disciplina del prelievo venatorio (almeno come si è constatato con la presentazione di emendamenti in Commissione). D'altro canto, non trovo ragionevole rimproverarsi il fatto di aver affrontato anche temi urgenti e rilevanti, quali l'adeguamento alla disciplina comunitaria comunitaria di servizi pubblici locali di rilevanza economica e la difesa del *made in Italy* o del prodotto nostrano, a cagione della scarsa attinenza di questi con altri argomenti trattati. Il Gruppo della Lega Nord ha ha optato per l'atteggiamento costruttivo, per il senso di responsabilità di fronte all'atto dovuto, agli obblighi impellenti che ci derivano da atti normativi comunitari e dalle sentenze della Corte di giustizia, anche entrando nel merito di questioni o meglio di una questione per noi controversa. Per la premura che ci muove nei confronti della nostra gente e del territorio, infatti, non nascondiamo di nutrire perplessità sugli effetti che le nuove regole potrebbero produrre in fatto di gestione dei servizi pubblici locali. Teniamo a sottolineare che in molte realtà padane sono presenti società erogatrici di servizi indispensabili, dalla fornitura dell'acqua potabile al gas, le quali offrono una condizione pienamente virtuosa secondo una logica di preminenza dell'interesse collettivo rispetto al mero profitto. Ebbene, vorremmo poter escludere che in un periodo di crisi, quando la produzione si contrae e il rischio di impresa lievita, qualcuno possa progettare di rifarsi lucrando sui beni primari. Crediamo, dunque, che occorra una valutazione approfondita della disciplina dei servizi pubblici locali, anche nell'ottica di prevedere maggiori garanzie per il cittadino. sollecitudine di tutela del consumatore e del produttore è risolutamente affermata in altro punto del provvedimento: quell'articolo 16 che finalmente definisce senza ambiguità i requisiti indispensabili del *made in Italy* e del prodotto italiano, prevedendo per falsificatori e contravventori un drastico inasprimento delle pene e pesanti sanzioni pecuniarie. In tutta sincerità, colleghi senatori, credo che le critiche di chi storce il naso lamentando l'eterogeneità del provvedimento saranno abbondantemente compensate dal sorriso di tanti lavoratori. Penso anche agli addetti del settore tessile, a cui ci siamo particolarmente riferiti, che forse potranno tirare un respiro di sollievo davanti all'argine posto contro la dilagante contraffazione che si traduce in perdita di capitali ingenti e posti di lavoro. Riflessioni, questa ancor più delle precedenti, che inducono ad esprimere una valutazione nel complesso positiva sulla conversione in legge di un decreto-legge considerato come un atto dovuto, scaturito da obblighi comunitari, ma che, credo, ci ha offerto l'opportunità di fare di necessità virtù. *(PD)*. Signora Presidente, signor Ministro, colleghi, affinché non sia solo un dibattito tra specialisti tenterò di sollevare tre questioni che riguardano questo argomento e che, in parte, sono state già evidenziate prima, anche dal collega che mi ha preceduto. Innanzitutto mi sembra consolidato in questa Aula il giudizio su questo decreto-legge: stiamo parlando, sostanzialmente, di una di una "paracomunitaria", e questo in presenza di una legge comunitaria che sta terminando il suo *iter*, nel senso che è stata già approvata dalla Camera dei deputati e che, come opportunamente viene specificato nella relazione, a breve sarà anche al Senato. Quindi, in pratica, ci troviamo di fronte ad una legge che ripercorre il modo di essere di una legge comunitaria. Ma si tratta di un decreto-legge perché si ritiene vi siano necessità e urgenza rispetto

che l'attuale Ministero - gliene do atto - sta cercando di ridurre, ma con mezzi minori di quelli precedenti perché c'è un problema di relazione tra questo Governo e l'Unione europea. Ma, comunque,

bisognerebbe rivedere il fatto che non sia affidato al settore agroalimentare il controllo degli alimenti piuttosto che alla Sanità, ma è una vecchia questione che rimarrà materia sulla quale dibattere. In ogni caso, viene affidato di fatto alla Sanità militare

Abbiamo presentato degli emendamenti costruttivi; abbiamo preso atto che, a nostro avviso, non c'era necessità e urgenza, ma che poteva essere aperto comunque un dibattito su alcuni di questi argomenti.

*(PdL)*. Signora Presidente, signor Ministro, il provvedimento in esame si inscrive in una prassi che si è affermata negli ultimi anni e che vede il recepimento della normativa comunitaria ripartito in due grandi moduli di intervento: la legge comunitaria annuale e i decreti-legge cosiddetti antinfrazioni.

infatti, necessari per dare una risposta ad una duplice esigenza: vi è, da un lato, quella di una risposta al mercato che chiede alle istituzioni nazionali un pronto recepimento delle norme comunitarie, oramai parte integrante della vita di tutti i giorni e parte essenziale della vita degli affari dall'altro, quella di una risposta alle istituzioni comunitarie che ci impongono, con ferma determinazione, un adeguamento corretto e nei termini, al fine di permettere quell'integrazione fra ordinamenti che è la base stessa della costruzione europea. Questo è il motivo per cui alla legge comunitaria si è affiancato lo strumento delle misure urgenti. Ciò naturalmente non toglie che tale modalità di adeguamento alla normativa comunitaria debba essere limitato a ciò che è assolutamente necessario, per permettere alla legge comunitaria di trattare le rilevanti questioni connesse all'ingresso delle norme europee nel nostro ordinamento con l'approfondimento necessario.

Tale disposizione consente l'emanazione di provvedimenti normativi, anche urgenti, per far fronte ad atti normativi o a sentenze che comportino obblighi statali di adeguamento, allorquando la scadenza di tali obblighi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso. Poiché le disposizioni del decreto-legge attengono ad obblighi comunitari già scaduti e posto che l'*iter* di approvazione della legge comunitaria per l'anno 2009 si è concluso alla Camera dei deputati ma non è ancora iniziato al Senato della Repubblica, i presupposti descritti dall'articolo 10

introduce misure urgenti per la promozione dell'ambientalizzazione delle imprese in armonia con le direttive europee in tema di riduzione delle emissioni e prevede impegni di riduzione differenziati delle emissioni di C02 da Paese a Paese.

fra la mitigazione delle cause di tali cambiamenti e l'adattamento agli effetti da essi prodotti, trasformando la necessità di agire in un motore di sviluppo economico e sociale. Per questo è necessario intervenire favorendo misure alternative al trasporto su gomma.

tra i traffici di merci su rotaia in area continentale, che attraversano l'arco alpino, e i traffici di merci tramite cabotaggio nel Mediterraneo. A mio giudizio è necessario agevolare il trasporto fluviale ottimizzando l'efficienza delle infrastrutture esistenti e favorendo l'intermodalità degli elementi della

che mira a sanare la procedura di infrazione n. 4145/2008 di costituzione in mora, ex articolo 226 del Trattato CE, mediante la quale la Commissione europea ha evidenziato alcuni punti critici del regime fiscale applicato in Italia ai proventi derivanti dalle partecipazioni ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie (i cosiddetti fondi non armonizzati). Secondo la Commissione europea, il regime fiscale di tali fondi presenta dubbi di compatibilità con i principi del diritto comunitario relativi alla libera circolazione dei capitali all'interno dell'Unione europea garantiti dall'articolo 56 del Trattato CE e dall'articolo 40 dell'Accordo sullo La procedura di infrazione concerne il disallineamento tra il trattamento fiscale dei proventi conseguiti da persone fisiche non aventi la qualità di imprenditore aventi la residenza in Italia, derivanti dalla partecipazione a fondi mobiliari non armonizzati di diritto estero per la parte qualificabile come reddito di capitale, ed il trattamento fiscale dei proventi derivanti da fondi mobiliari non armonizzati italiani, sempre conseguiti da persone fisiche non aventi la qualità di imprenditore ed aventi la residenza in Italia. Con l'articolo 14 si cerca di porre rimedio a tale discrasia. Tuttavia il decreto-legge sembra accentuare il trattamento fiscale differenziato che esiste tra le varie tipologie di organismi di investimento collettivo del risparmio negoziate in Italia. Italia. In particolare, i fondi di diritto italiano sono tassati con aliquota sostitutiva del 12,50 per cento sul risultato di gestione maturato nell'anno di riferimento, mentre i fondi esteri sono tassati con aliquota sostitutiva del 12,50 per cento sulla differenza tra il valore di riscatto il valore di sottoscrizione o acquisto. Appare quindi opportuno che tale differenziazione venga eliminata, anche in considerazione dell'operatività del principio di parità di trattamento di ispirazione comunitaria. Di conseguenza, o l'articolo 14 deve essere soppresso rimandando rimandando la disciplina della complessa materia ad un provvedimento *ad hoc,* oppure dobbiamo inserire la previsione che per i fondi mobiliari chiusi si passi dalla tassazione sul maturato a quella sul realizzato.

Stato il legittimamente concessi alle ex municipalizzate. Non è un *unicum* nel panorama italiano in quanto esiste un altro filone di aiuti di Stato illegittimamente concessi. In relazione a questo c'è una importante decisione della Corte costituzionale, con la quale sono stati ricordati alcuni principi della giurisprudenza comunitaria in materia di azioni di recupero di aiuti illegittimi. In realtà, il centro del problema per la Corte costituzionale aiuti illegittimi. In realtà, il centro del problema per la Corte costituzionale riguarda il termine breve di prescrizione. A mio avviso, andrebbe approfondito questo passaggio al fine di verificare la possibilità di prevedere un termine breve di prescrizione per queste azioni, magari modellato sulla falsariga del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità extracontrattuale dei singoli verso le istituzioni della comunità. Concludendo, signora Presidente, Ministro, questo provvedimento dimostra che, come abbiamo detto all'inizio, le norme comunitarie sono ormai parte integrante della vita di tutti i giorni

l'incisività dell'azione dei parlamentari, in particolare quella operata in Senato, nella fase ascendente delle direttive.

- specificamente dalla Provincia autonoma di Trento - dove l'applicazione degli obblighi comunitari è stata rigorosa al punto da portare a discriminazioni a rovescio nei confronti di lavoratori italiani, penalizzati - guarda un po' - rispetto a lavoratori provenienti da altri Stati membri.

cui deve conseguire la fase della libera circolazione delle professioni e rispettivi riconoscimenti delle tali, fino ad arrivare a quella che abbiamo conosciuto, l'integrazione monetaria, cioè un contesto

questo è l'*iter*, questo sarà il futuro della nostra comunità. Il fine comunque che ci siamo prefissati è di avere una grande area di libero scambio, di reciproci reciproci riconoscimenti, finalizzata ad avere innanzitutto un libero mercato: ciò sta a significare che con la libera concorrenza i cittadini avrebbero avuto le massime garanzie,

sintetizzare, è questa grande opportunità, un mezzo che ci potrebbe consentire di raggiungere questo grande fine.

cercando di aggirare gli obblighi comunitari. Si parla di regole, o meglio, di norme protezionistiche, che non si possono più adottare, però vediamo in quante occasioni gli Stati tentano - è giusto o, almeno, si può capire - di aiutare la propria economia, mettendo un po' un freno a questa grande e libera concorrenza europea. Con riguardo agli aiuti di Stato, ogni Stato si trova sempre sul crinale: fa delle operazioni di aiuto e di sostegno dell'economia e delle imprese interne a volte scavalcando questa piccola, labile linea di demarcazione tra ciò che è possibile e ciò che va contro le va contro le normative europee. Tutto ciò è comprensibile, giusto o sbagliato che sia. Adesso entriamo nello specifico della di circolazione delle professioni e dei riconoscimenti reciproci delle rispettive professioni. Non c'è dubbio che non siamo in presenza di un'integrazione completa: le formazioni professionali non sono identiche in tutta Europa.

In Spagna l'avvocato non deve superare alcun tipo di esame di Stato: una volta laureatosi in giurisprudenza, si iscrive ad un albo, esercita, fa un tirocinio e svolge la professione di avvocato. Non c'è dubbio che se dobbiamo riconoscere la professione di avvocato non possiamo pretendere che l'avvocato spagnolo entrando in Italia si sottoponga ad una successiva ulteriore verifica secondo i parametri italiani. E ciò vale per tante altre professioni. alla professione del maestro di sci. Ogni Stato abilita a questo esercizio professionale con dei corsi, con dei *curricula* che sono diversi (e probabilmente quelli italiani sono fra i più lunghi, più rigorosi e meticolosi e forse danno una preparazione migliore rispetto a tanti altri Stati).

che il cittadino italiano con lo stesso medesimo brevetto, per il semplice fatto che non è un cittadino di Stato membro ma è cittadino italiano, non la può esercitare e si deve sottoporre a un ulteriore corso, un prolungamento della preparazione e a una verifica finale, cosa che non è richiesta al cittadino di uno Stato membro, al cittadino non italiano.

siamo di fronte a un decreto‑legge che si riferisce alle disposizioni relative all'attuazione di obblighi comunitari. Questa mattina, nelle questioni pregiudiziali presentate, i colleghi del mio Gruppo e degli altri Gruppi di opposizione hanno sostenuto che vi sono molte norme che non hanno nulla a che vedere con l'attuazione di obblighi comunitari e che pertanto sono state inserite surrettiziamente, riproponendo una prassi che è stata più volte denunciata, anche dalla Presidenza della Repubblica, come assolutamente inaccettabile dal punto di vista dell'attuazione dei principi costituzionali. La prova evidente di ciò è l'emendamento,

perché tutti ricordiamo quanto sia stata forte la discussione in quest'Aula e alla Camera sulla legge relativa al federalismo fiscale, quanto sia stato importante il confronto svolto in quell'occasione e il contributo che le opposizioni hanno dato al provvedimento, che ha consentito di arrivare ad un voto di astensione da parte del Gruppo del Partito Democratico. Tale astensione era motivata, tra l'altro, anche da una diversa scansione temporale prevista, al comma 6 dell'articolo 2, dei decreti legislativi attuativi.

il quale il Governo avrebbe provveduto all'attuazione della delega. Da parte nostra, in modo particolare, si è insistito per avere una successione temporale più definita. Il comma 6 stabiliva che entro 12 mesi doveva essere altro decreto legislativo doveva essere approvato in relazione ai costi e ai fabbisogni standard e, contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo,

struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse, ossia il tema dei conti. Una delle critiche fondamentali che abbiamo avanzato nel corso della nostra discussione è stata circa l'impossibilità di approvare una legge sul federalismo fiscale senza le simulazioni in termini di effetti finanziari, indispensabili per capire dove si vuole andare a parare. Quindi, uno dei motivi per i quali abbiamo offerto il nostro contributo, arrivando anche ad un voto di astensione su quel provvedimento, era esattamente questo: poiché il Governo, attraverso il ministro Tremonti, più volte ci ha detto che era impossibile provvedere a simulare gli effetti della legge prima di averla approvata, noi abbiamo in qualche modo acceduto a questa idea, abbiamo rinunciato alla nostra proposta originaria, quella di richiedere una simulazione finanziaria contestualmente alla discussione in Aula della legge e, quindi, abbiamo approvato, insieme alla maggioranza, l'idea di demandare tutto al primo schema di decreto legislativo.

si parla di un decreto legislativo sull'armonizzazione dei bilanci pubblici che dovrebbe essere emanato dal Governo tra dicembre e gennaio e, quindi, definitivamente approvato entro marzo o aprile, e ora, invece, si rinvia tutto di due, tre mesi.

ci allarma moltissimo perché riteniamo che a questa altre ne potranno seguire sempre nella stessa direzione. Mi rivolgo quindi in modo particolare al Gruppo della Lega Nord, che attribuisce al tema del federalismo fiscale un'importanza decisiva anche per l'andamento di questa legislatura. Cari colleghi, se io fosse in voi, sarei molto preoccupato per questa piccola modifica, apparentemente piccola ma, in realtà, molto significativa di un atteggiamento, quello del Ministero dell'economia che, come è stato durante la discussione della legge sul federalismo fiscale, ancora una volta denota un disimpegno completo da questo tema. Sappiate che nel corso della discussione sul decreto‑legge in esame noi continueremo a sostenere questo argomento perché lo troviamo davvero emblematico del modo con il quale da una parte si annunciano grandi riforme federaliste e dall'altra poi le si calpestano nei fatti.

Senato; quel nostro voto di astensione, infatti, era legato, tra le altre cose, anche a questa norma. Pertanto, noi chiediamo che venga ripristinato il testo originario, che venga cancellato il comma 3 del nuovo articolo 19-*bis* del decreto, in primo luogo perché non ha nulla a che vedere con le questioni di cui stiamo parlando e perché poi nella sostanza è profondamente lesivo della possibilità di attuare davvero il federalismo fiscale che noi vogliamo ma, a quanto pare, la maggioranza e il Governo molto di meno. finestra"). Onorevoli colleghi, sono presenti in tribuna gli alfieri del lavoro. Desidero esprimere a tutti loro e agli studenti del collegio di eccellenza dei cavalieri del lavoro, del quale alcuni fanno parte, i rallegramenti dell'Assemblea del Senato per i brillanti risultati conseguiti nel loro percorso scolastico, che premia l'impegno e la determinazione nello studio, di cui siamo tutti orgogliosi.

Preme innanzitutto rilevare l'inadeguatezza dello strumento utilizzato. Si è scelto di far confluire in un decreto *omnibus* temi di notevole rilevanza non avvinti da alcun nesso di pertinenza. A mero titolo esemplificativo, non già esaustivo, si disciplinano nello stesso provvedimento legislativo temi quali le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, la definizione del prodotto *made in Italy*, del prodotto interamente italiano, il regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari esteri non armonizzati. Fittiziamente, nell'illustrazione del provvedimento *de quo* si è affermato che il suo fondamento è da ravvisarsi nella necessità di adempiere ad obblighi comunitari giunti a scadenza, al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 117, comma primo, della Costituzione. La Commissione europea, a causa del ritardo o del non corretto recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento nazionale, ha dato infatti avvio a numerose procedure d'infrazione nei confronti dello Stato italiano. Con il suddetto decreto si sarebbe dovuto porre rimedio alle esatte censure mosse dalla Commissione europea, al fine di evitare un aggravio di oneri a carico dello Stato, derivanti da possibili sentenze di condanna a pene pecuniarie da parte della Corte di giustizia o derivanti da contenzioso interno, ma così non è. Ebbene, preso atto degli emendamenti depositati presso la Commissione affari costituzionali, ci si interroga sull'ammissibilità di emendamenti del tutto estranei all'oggetto della discussione, in spregio dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento. Le medesime perplessità sono sorte persino ad esponenti del Governo durante l'esame del provvedimento in sede consultiva nell'8a Commissione, che hanno constatato come gli emendamenti proposti ed accolti non appaiono necessitati dall'esigenza di prevenire il contenzioso con la Commissione europea ma ai quali sono semmai sottese finalità misconosciute. All'uopo, con un emendamento, il 3.0.5, presentato dal relatore Malan, si è persino inciso in materia di federalismo infrastrutturale. Sostanzialmente si vorrebbero limitare le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore dei soggetti di diritto pubblico appositamente costituiti in forma societaria e partecipati dalle Regioni e dall'ANAS alla sola realizzazione di infrastrutture autostradali che ricadano esclusivamente nel territorio di interesse regionale. Con una circonlocuzione chiara si escludono le Regioni dalla gestione delle concessioni autostradali; quasi nessuna infrastruttura autostradale è, infatti, di esclusivo interesse regionale. Il federalismo infrastrutturale fu voluto dall'allora ministro delle infrastrutture, onorevole Antonio Di Pietro, al fine di conferire alle Regioni un ruolo di attrici nel procedimento di aggiudicazione delle concessioni autostradali e non già di mere spettatrici dell'operato dell'ANAS ed era volto a far sì che le entrate legate ai pedaggi, per lo più provenienti dalla popolazione residente sul territorio, al netto degli investimenti e delle spese, rimanessero nel territorio, così da costituire una fonte cui attingere per la realizzazione di ulteriori infrastrutture. Cari colleghi, il federalismo dell'attuale Governo vorrei chiamarlo «federalismo del gambero». Spesso ho rinunciato ad una polemica, a volte fin troppo facile, offrendo leale collaborazione per realizzare obiettivi essenziali per il nostro Paese, ma oggi non posso tacere dinanzi a tutto questo. Nell'attesa del federalismo che verrà si distrugge quel che già c'è. Si escludono le Regioni dalla gestione delle concessioni autostradali, con grave detrimento sia per la realizzazione delle medesime infrastrutture autostradali che per le finanze delle Regioni, già ampiamente decurtate. Leggendo questo articolo sembra esser ritornati all'epoca medioevale, era la massima valorizzazione dei feudatari, più o meno nuovi, a detrimento del popolo al quale, è bene rammentarlo, la Carta costituzionale all'articolo 1 attribuisce la vera sovranità. Ai cittadini, in posizione servente rispetto ad essi, si affiancano poi gli enti locali, ex articolo 5 della Costituzione, che, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale, ne amministrano i servizi.

se arriverà un nuovo Mosè capace, tornato dalla preghiera e scoperto che il proprio popolo è tornato a venerare un Dio pagano scordandosi della terra promessa, di scuotere il Governo. Temo di no, pertanto, in questa sede mi faccio portatore dei diritti dei cittadini a nome del Gruppo Italia dei Valori. L'esercizio dei poteri e delle funzioni di soggetto concedente ed aggiudicatario delle concessioni autostradali devono rimanere agli enti locali e non al mercato, a nuovi signori, e men che mai a società quotate totalmente private, ossia agli investitori, che, peggio degli operatori di epoca feudale, passati da logiche mutualistiche a quelle commerciali ed imprenditoriali, sono infine approdati con i cosiddetti *hedge fund* a soldi moltiplicatori di soldi. Il Governo propone, nell'ambito della conversione di un decreto-legge recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle non è volto ad eliminare alcun contrasto tra la normativa comunitaria, *sub specie* «tutela della libera concorrenza», e la peculiare disciplina prevista dai commi 289 e 290 dell'articolo 2 In conclusione, i fatti palesano una forte discrasia tra ciò che in astratto si declama e ciò che in concreto si realizza. Il Governo sembra gettare la maschera e mostrare la sua ritrosia verso il federalismo che, a suo tempo, ha rappresentato un cavallo di battaglia agevole da cavalcare, ma che ad oggi sembra apparire scomodo e non meritevole di rispetto. Un ultimo cenno vorrei rivolgerlo alla modifica che viene apportata con il provvedimento *de quo* alla disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica. Appare evidente la spinta del Governo verso le privatizzazioni, in linea con la strategia di progressiva liberalizzazione dei servizi concordata a Marrakech in sede di WTO nel 1994 e ripresa nella Strategia di Lisbona nel 2000, ma che, ad oggi, a seguito delle numerose criticità emerse, è in corso di revisione. In questa sede non entrerò nel merito della riformulazione dell'articolo 23-*bis* della legge 6 agosto 2008, n. 133, ma non posso omettere di porre l'attenzione sul servizio idrico. L'inclusione di questo settore nella disciplina generale dei servizi di interesse economico non è tollerabile. L'acqua è un bene comune che deve necessariamente essere ripubblicizzato. il ministro francese François Fillon ha sottolineato la necessità della riaffermazione del ruolo dello Stato nel settore dei servizi pubblici. Lo stesso Benedetto XVI, nella sua recente enciclica *Caritas in veritate*, ha affermato che «l'accesso all'acqua è un diritto universale di tutti gli esseri umani senza distinzione e discriminazioni». Tutto questo è legato al diritto primario alla vita. L'acqua è vita! È intollerabile che la gestione del servizio idrico venga assimilata a quella relativa ai rifiuti. Si tratta della mercificazione di una risorsa essenziale. Non si può assistere silenti innanzi ad un Governo che si fa paladino dei potentati economico-finanziari. La forza del mercato sembra spazzar via ogni istanza egualitarista. Si afferma il falso quando si dice che il servizio idrico integrato deve ricadere nella disciplina prevista per i servizi pubblici di rilevanza economica.

in materia di determinazione dei programmi e dei controlli. Nel modificare la disciplina dei servizi pubblici locali si è poi omesso di introdurre modifiche importanti quali il principio di separazione proprietaria tra le imprese che gestiscono la rete e le imprese che erogano il servizio.

mi permetto di richiamare uno di questi casi che, fino a qualche ora fa, ha provocato, non dico la messa a ferro e a fuoco, ma comunque grandi proteste in Sardegna, con un semiblocco dell'aeroporto di Cagliari e l'invasione da parte dei lavoratori del settore alluminio dell'ALCOA del Consiglio regionale e della Regione autonoma della Sardegna. Si tratta di una procedura di infrazione aperta sin dal 2006 2006 riguardante le tariffe energetiche che consentono nel nostro Paese, sia in Veneto che in Sardegna, il mantenimento di questo tipo di produzione;

ha evitato molto accuratamente di venire in Sardegna a discutere con i lavoratori di questi problemi, pur avendo annunciato una sua visita: si è dato malato seppure imperversa nelle agenzie di stampa con dichiarazioni sul PdL siciliano; evidentemente vi sono problemi di cui il Ministro dello sviluppo economico può permettersi di non curarsi! Egli ha affermato in quest'Aula e in atti pubblici e di indirizzo derivanti dall'operato del Parlamento che la questione era chiusa e che aveva negoziato con l'Unione europea la soluzione del problema delle tariffe energetiche consentendo la permanenza nel nostro Paese delle produzioni di alluminio, un metallo particolare fortemente orientato alle produzioni tecnologiche. dalla multinazionale americana che produce in Italia l'alluminio - che ciò non sia vero e che l'Unione europea, nonostante gli atti promessi dal Governo, mantenuti dal Parlamento e attuati sempre dal Governo nelle settimane scorse, si stia accingendo a chiudere negativamente la procedura di infrazione con oneri di restituzione che vanno dai 200 ai 600 milioni di euro e che cancellerebbero questo settore industriale dal panorama produttivo del Paese. Mi chiedo, al di là del profilo di ordine pubblico (si tratta di 2.000 lavoratori che finirebbero la loro attività con la chiusura delle aziende, già annunciata per il 17 novembre quale sia l'attenzione del Governo a casi come questi, che non riguardano etichettature né profili secondari

Signora Presidente, vorrei appuntare la mia attenzione sulle norme riguardanti i temi energetici

Ovviamente tutti sappiamo che la Corte di giustizia ci ha più volte sanzionato per il ritardo con cui l'Italia si adegua alla normativa europea e quindi sono state avviate alcune procedure di infrazione. In questo caso, la motivazione dell'intervento non è tanto da rinvenirsi in queste procedure di infrazione, quanto nel mancato coordinamento tra l'articolo 27 della recentissima

all'articolo 4, per i commi 3, 4 e 5, che recano misure per la promozione dell'ambientalizzazione delle imprese. In questa parte della norma a nostro parere nulla si dice circa gli straordinari motivi di necessità e urgenza che suggerirebbero l'inserimento di queste disposizioni in questo provvedimento, anche alla luce del fatto che esse contengono una sorta di delega in bianco ai Ministri dell'ambiente e dello sviluppo. Non è la prima volta che il Gruppo dell'Italia dei Valori denuncia come in molti provvedimenti esaminati dall'Aula vi siano deleghe in bianco ai Ministeri, di cui poi non si ha più il controllo. il controllo. In particolare, si prevede che con decreto ministeriale siano approvate specifiche linee guida recanti, anche in questo caso, non meglio precisati criteri e parametri per la promozione degli investimenti in innovazioni tecnologiche. Queste ultime - è detto - devono essere finalizzate alla protezione dell'ambiente, alla riduzione delle emissioni, alla riduzione del consumo delle risorse naturali e all'incremento dell'efficienza energetica. Si tratta, teoricamente, di una lodevole finalità. Tuttavia - questo è un aspetto che voglio evidenziare - l'unico ancoraggio previsto appare il rispetto dei «valori minimi previsti dalle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili» di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 59 del 2009.

«l'attribuzione di coefficienti e caratteristiche di qualità ambientale ai predetti impianti in funzione del rispetto degli anzidetti criteri e parametri».

ancora, poiché si parla di raffinerie di petrolio, di centrali termiche, di impianti di combustione con potenza superiore ai 300 megawatt, acciaierie e impianti chimici di notevoli dimensioni, occorrerebbe - a nostro parere - quanto meno esplicitare e chiarire una serie di aspetti che vado ad elencare. Innanzitutto, occorrerebbe esplicitare l'esatta rispondenza alle norme, ai limiti e ai parametri comunitari di tutela ambientale, sanitaria e di

di coefficienti sono limitati agli impianti che dimostrano di aver rispettato in passato e di poter rispettare in futuro la normativa nazionale e comunitaria vigente, avendo adottato le migliori tecnologie disponibili. escludere ogni pur remota e residuale possibilità di individuare coefficienti, limiti, o parametri meno cautelativi rispetto a quelli esistenti, con particolare riferimento al tema delle emissioni. Queste cautele, che ci paiono elementari, elementari, non sarebbero di per sé assolutamente indispensabili se la vaghezza della formulazione non ci lasciasse presagire o temere possibili inconvenienti in sede applicativa; ci sembrano tanto più necessarie ove si pensi che all'individuazione dei coefficienti e delle caratteristiche di qualità ambientale degli impianti, discrezionalmente rimessa a quel decreto ministeriale di cui ho parlato prima, prima, consegue il dimezzamento dei termini istruttori previsti dal decreto legislativo n. 59 del 2005. Lo stesso vale per gli impianti di nuova realizzazione soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, che hanno richiesto tale autorizzazione dopo l'entrata in vigore del decreto correttivo del codice ambientale, ossia il decreto legislativo n. 4 del 2008.

la necessità di adempiere ad obblighi comunitari ha rappresentato per il settore del mondo agricolo un'opportunità che, sia il Ministro dell'agricoltura sia questo Governo, sono stati brillantemente in grado di cogliere, intervenendo in maniera puntuale su alcuni temi di assoluta attualità e di rilevanza per il mondo agricolo In primo luogo, le norme a tutela del *made in Italy*, nel cui ambito si è data la giusta collocazione ed importanza ai prodotti agroalimentari

Al riguardo, non possiamo assolutamente dimenticare che l'industria alimentare è il secondo comparto dell'industria manifatturiera del nostro Paese e che l'intero settore agroalimentare in questo periodo sta soffrendo una crisi economica rilevante. Tutto questo ha pienamente confermato il suo carattere anticiclico, che nel suo complesso ha recato importanti benefici all'intero sistema economico nazionale, segnando anche alcuni importanti risultati, primo tra tutti,

Ancora oggi, ancora una volta, è l'agricoltura il settore che ci permetterà di combattere questa crisi. E non può che essere così in un paese fisiologicamente privo di materie prime,

Dobbiamo essere coscienti del fatto che senza l'agricoltura molto probabilmente, anzi sicuramente, non ci sarebbe neanche economia. Le nostre proposte sono finalizzate

preventivamente approvate in quest'Aula e attualmente sono all'esame della Camera dei deputati, norme riguardanti il provvedimento in materia di etichettatura

un ulteriore stanziamento a favore delle attività di controllo della contraffazione. Tali attività sono indispensabili visti i dati in nostro possesso, che ci dicono

Di uguale importanza, attualità e tempestività sono da considerare le disposizioni in favore dei produttori di latte, che oggi risultano in regola con il regime delle quote e che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008.

n. 119 del 2003 con le nuove realtà normative e produttive nate anche dalla modifica della PAC, vengono fornite oggi con questo provvedimento pronte risposte ad un settore che ormai da troppo tempo vive una situazione

abbiamo portato a casa anche alcune misure che, unitamente a quelle proposte, riusciranno a dare liquidità alle imprese, ai nostri giovani;

Credo che sia giusto anche sottolineare la grande tempestività con cui il Governo è riuscito a porre in essere tutte le condizioni necessarie affinché possa essere garantita l'esecuzione anche per quanto riguarda il censimento dell'agricoltura,

evoluzione verso il biologico, verso l'agriturismo, verso forme di artigianato legate al mondo della produzione agricola. Tutto questo al fine di intervenire con nuove e più adeguate strategie,

accettare il contributo, anche se critico, che l'opposizione dà - e lo fa nell'interesse generale del Paese - è il segno di una cultura politica matura. Una cultura politica che sola può garantire che il nostro Paese abbia il giusto peso politico nell'Unione europea. È questo a mio modo di vedere l'obiettivo che deve impegnare tutti quanti, maggioranza e opposizione, penso che per questo c'è un urgente bisogno di cominciare a giocare come sistema Paese nelle sedi europee e perché ciò sia possibile questo sistema Paese deve cominciare a funzionare prima di tutto in Italia, a partire dal suo Parlamento,

per porre un argine al fenomeno delle infrazioni, per recuperare il pregresso ma anche perché il recepimento sia concreto, materiale e non mero adempimento formale del diritto comunitario. Non sarebbe questa condivisione cosa da poco, caro Ministro, nell'attuale clima politico interno, né sarebbe la prima volta che l'Europa agendo da vincolo esterno diventa la leva del cambiamento positivo capace di dare forza ed autorevolezza al nostro Paese. Per quanto mi riguarda, sono tre gli ordini di questioni che palesemente fanno di questo decreto contemporaneamente uno scandalo legislativo e un'offesa al lavoro serio che viene svolto nelle Commissioni. Ai commenti dei miei colleghi di Gruppo su questi tre ordini di questioni, voglio aggiungere un ragionamento più attinente al nostro vivere e stare in Europa. innanzitutto una questione di metodo: laddove ciascun Paese membro dell'Unione europea ha adeguato o lo sta facendo il *modus operandi* del proprio Parlamento per adeguarsi alle norme introdotte dal Trattato di Lisbona e sottolineare così con tali modifiche operative la propria presenza sullo scenario europeo rendendola più incisiva, il Senato italiano non solo non riesce ad avviare la discussione su una modifica del Regolamento - le proposte di modifica in tal da quella presentata dalla Commissione politiche dell'Unione europea con l'accordo di tutti Gruppi politici - ma crea al contempo di fatto le condizioni per un peggioramento della situazione. L'uso indiscriminato di decreti contenitori onnicomprensivi, veri calderoni, è un'arma contro il Parlamento che, a mio avviso, va spuntata per ricondurre il dibattito alle regole democratiche e recepire il contributo di tutti. In quanto al secondo ordine di questioni, è già stato detto - non voglio per questo entrare nel merito - che il decreto di cui oggi discutiamo ha una scarsissima corrispondenza tra il titolo e il suo contenuto. La scarsissima corrispondenza è ulteriormente peggiorata dai numerosi emendamenti presentati dalla maggioranza e dal relatore, molti dei quali di chiara provenienza governativa. emendamenti che in alcuni casi configurano un aggravamento della situazione di infrazione e che in altri servono solo ad aggirare obblighi comunitari o ad allentarne i criteri; negli altri casi nulla hanno a che vedere con la materia che qui dovremmo trattare. Il recepimento degli obblighi comunitari e il conseguente risanamento delle procedure di infrazione si configura da noi come mero adempimento formale, anziché come strumento per il rinnovamento del sistema Paese, che ha la sua base nel partenariato istituzionale e non in quello politico. I ritardi che accumuliamo, come ci è stato confermato nelle numerose audizioni che la Commissione politiche dell'Unione europea ha svolto sul tema dell'utilizzo dei fondi comunitari e dell'adempimento degli obblighi conseguenti, ha come prima ragione l'assenza di un modello di pianificazione dello sviluppo imperniato su uno Stato centrale che realizza indipendentemente dalla compagine politica del momento. Abbiamo perciò bisogno di un forte impegno politico, affinché la programmazione non resti esercizio di stile e di allocazione di risorse e l'attuazione si riduca a prassi burocratico-amministrativa

Stiamo parlando di oggi, caro Ministro. Sarebbe bene, allora, avere chiaro che in tema di attuazione del principio cardine dell'addizionalità e della sussidiarietà la Commissione europea può, in relazione al grado di inadempimento di tale obblighi, procedere ad una rettifica finanziaria, sopprimendo la totalità o una parte del contributo concesso ad uno Stato a titolo di fondi strutturali. Dico questo, cari colleghi, non certo per tediarvi con dettagli tecnici, che tanto dettagli non sono, ma per ribadire che non basta l'esercizio dell'adempimento così come LA mera allocazione di risorse; dobbiamo alzare il tiro soprattutto rispetto alla qualità del nostro legiferare e programmare. Per mutare la rotta occorre perciò una riflessione di ampio respiro sul nostro europeismo ed una maggiore condivisione sugli obiettivi da raggiungere. Valga per tutti il già citato esempio dell'articolo 15, la famosa direttiva servizi, che da solo vale come esempio di quanto sto affermando; ma non vanno dimenticate neppure le modifiche proposte alla legge comunitaria 2008 a distanza di pochissimi mesi dalla il non voler sanare le infrazioni relative alla direttiva sulle frequenze televisive, mentre si approfitta di questo decreto per liberalizzare ulteriormente pratiche commerciali pubblicitarie. Terzo ed ultimo ordine di questione, signor Presidente. Il dibattito su questo decreto-legge è un'occasione che noi - ma come abbiamo sentito nel corso del dibattito anche molti esponenti della maggioranza non vogliamo perdere per evitare di mettere ancora più in ginocchio i Comuni, per non prendere in giro gli italiani che hanno creduto nel federalismo fiscale, per coerenza ed onestà e soprattutto per non svuotare dei suoi poteri la Commissione politiche dell'Unione europea. inoltre, come troppo spesso sta accadendo di occuparci con i soldi dei contribuenti di interessi molto particolari, a detrimento dell'interesse comune dell'Italia e dell'Unione europea. Signor Presidente, questa è la nostra convinzione e credo debba essere il nostro costante punto di riferimento, soprattutto ora che si torna a parlare di rilancio del processo di integrazione politica dell'Unione per porre fine all'incertezza decisionale da più parti denunciata, anche da questo Governo. Ciò significa per noi più responsabilità non solo per chi ha funzioni di Governo, ma anche per chi sta all'opposizione. A questa sfida noi vogliamo corrispondere, nella chiarezza però e nella trasparenza delle posizioni, ridando vigore e forza al ruolo del Parlamento al fine di garantire partecipazione e condivisione del più grande ed originale progetto politico che l'unione di Stati e di popoli rappresenta. *(Applausi

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, credo che questo dibattito si sia sviluppato in Commissione, come pure in Aula, in modo assolutamente costruttivo e corretto. corretto. La collega Marinaro nell'intervento che mi ha preceduto invitava tutti noi ad una riflessione sul nostro modo di essere europei, sul nostro modo di vedere l'attuazione delle direttive comunitarie del processo di integrazione europea. Senza dubbio, l'Italia e gli italiani sono il Paese più europeista:

abbiamo ricevuto molte procedure di infrazione, siamo talvolta poco attenti alla difesa dei nostri interessi nazionali, diversamente da Paesi come la Francia e la Germania,

nelle maglie delle direttive dell'Unione europea di tutelare i nostri interessi nazionali. Alla luce di ciò, non riesco a capire però perché la polemica su questo provvedimento si sviluppi su quattro temi che ritengo fondamentali per gli interessi nazionali:

al provvedimento che consente di adottare bilanci omogenei alle Regioni e alle Province, al fine di creare i presupposti per la definizione del federalismo fiscale e l'individuazione dei costi standard. Sono quattro temi che vanno nella direzione della difesa degli interessi nazionali del Paese. Quanto ai servizi pubblici locali, è inutile continuare a dire che è una norma inconferente con questo disegno di legge; ha fatto bene il Governo ad inserire

questione del metodo *in house* per la gestione dei servizi pubblici dall'altro lato, perché vi era una notevole reazione alla possibilità di costruire queste società miste, pubbliche o private. Ma d'altro canto cosa facciamo, dopo tanti anni che abbiamo trasformato in società per azioni le municipalizzate, di fronte ad una verifica che vede oggi i nostri servizi pubblici tra i più arretrati d'Europa? Ci sono delle eccezioni sicuramente, però abbiamo dei limiti strutturali fortissimi, soprattutto con gli acquedotti. I dati che ci hanno presentato sono disastrosi: perdono il 40 per cento dell'acqua immessa negli acquedotti. Da decine di anni non si fanno più investimenti: o troviamo il modo per recuperare delle risorse attraverso il coinvolgimento dei privati o la situazione diventa emergenziale. Allora perché fare su questo tema ancora una battaglia ideologica? Non riesco proprio a capirlo. Lo l'articolo 16, relativo alla questione del *made in Italy*. Se avessimo avuto una norma come quella che abbiamo approvato, che ha avuto il consenso generale delle forze politiche, certamente avremmo evitato avremmo evitato situazioni catastrofiche in notevoli settori del nostro sistema industriale. Ne cito uno per tutti: per esempio abbiamo subìto in Italia una crisi nel settore di occhiali, che ci ha fatto perdere decine di migliaia di posti di lavoro perché viene falsificato il nostro modello: passano per *made in Italy* prodotti realizzati in Cina o nei Paesi dell'Estremo Oriente. Non era giusto introdurre norme di tutela della nostra produzione del nostro *made in Italy* fino in fondo? Abbiamo perso migliaia di dipendenti per non aver attivato questi meccanismi. credo che dobbiamo guardare alla sostanza e non metterci a parlare di questioni che appaiono ai più quasi burocratiche, cioè se un argomento è conferente o inconferente con questo provvedimento.

hanno fissato il termine delle concessioni autostradali agli attuali concessionari al 2040. Si stanno tutelando fino in fondo per gestire le infrastrutture, che sono per molti aspetti strategiche.

molti aspetti strategiche. Aver affrontato la questione del cosiddetto federalismo autostradale cercando di dare una soluzione a base regionale

Se non avessimo avuto questi meccanismi, per esempio nella realizzazione del Passante di Mestre, un nodo strategico fondamentale per il nostro Paese, esso non si sarebbe mai realizzato. Così pure devo ringraziare il Governo in questa occasione per aver assunto l'impegno di costituire una società mista tra la Regione Friuli-Venezia Giulia, Regione Veneto e ANAS per la gestione di quel nodo strategico, che è l'autostrada che da Venezia va verso Trieste e che è l'autostrada che ci collega

poter poi individuare i costi standard e quindi creare le premesse per la realizzazione del federalismo fiscale. Quindi, non c'è alcuna antitesi rispetto a ciò che abbiamo sostenuto in passato, nessuna voglia di rallentamento del processo riformatore del federalismo fiscale, ma tutti siamo d'accordo

due punti. Il primo è quello che riguarda i servizi pubblici locali. Come ho già detto durante la relazione introduttiva, sappiamo che sono state avanzate perplessità sullo strumento del decreto-legge per intervenire in questa materia. Constatiamo però che, grazie a questo intervento, stiamo arrivando ad un risultato che in qualche modo era stato auspicato da tutte le forze politiche, anche perché nelle scorse legislature già si era tentato di attuare una riforma in questo settore. I risultati saranno importanti per tutti: saranno positivi per gli utenti e per le amministrazioni degli enti territoriali, che potranno disporre di nuove risorse; saranno positivi sotto l'aspetto industriale, perché ci sarà un'apertura con la possibilità per nuove aziende - non soltanto quelle che, tutto sommato, hanno fruito

Molte altre critiche si sono appuntate sull'emendamento a mia firma riguardante la tutela della *privacy* delle telecomunicazioni. Vorrei sottolineare, e forse ci sarà occasione nel corso dell'esame del provvedimento, che non si tratta in nessun modo di dare via libera a coloro che abusano di questo strumento in modo fastidioso e molesto per i cittadini, ma di dare

sono argomenti di discussione e ci possono essere punti di vista diversi; non si tratta però assolutamente di un'apertura alle molestie telefoniche ma, al contrario, di approntare un sistema che tuteli davvero i cittadini da questa fastidiosa occorrenza.

innanzitutto permettetemi di ringraziare il presidente della Commissione Vizzini, il relatore Malan

Con l'articolo 15 riteniamo di compiere un passo fondamentale verso quello che, da ani, veniva visto come un desiderio che sarebbe rimasto inattuato, ovvero il riassetto del settore dei servizi pubblici locali.

Con l'articolo 19 abbiamo portato a definitiva soluzione uno dei problemi più annosi, che era penalizzante per il sistema delle municipalizzate. La scelta compiuta dal Governo è stata dolorosa, come sapete, ma ha consentito di chiudere una vicenda e un'infrazione che andava avanti da molti anni e rischiava di penalizzare proprio quelle aziende municipalizzate sane che costituiscono un importante tessuto connettivo in molte nostre città.

Si tratta di provvedimenti legislativi che risalgono a un'epoca precedente, al cosiddetto impegno Bersani, che ha legittimato affidamenti di questo tipo.

loro funzioni originarie, evitando che l'affidamento si possa tramutare in una sorta di speculazione. Su questo punto l'impegno del Governo sarà fermo e deciso sin dalle prossime settimane, con norme chiare e soprattutto con regole di assoluta trasparenza.

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione delle proposte 2.1000 e 19.1000. In ordine all'articolo 15, la Commissione esprime parere di semplice contrarietà per le seguenti ragioni: si formulano osservazioni critiche in relazione alle modalità applicative previste dalla disposizione, con particolare riferimento alla previsione del 31 dicembre 2012 quale data improrogabile entro la quale procedere alla riduzione della quota

connessi a una concentrazione temporale dell'offerta e ad un conseguente effetto di diminuzione dei valori di mercato delle quote in rilievo, risultando necessario sotto tale profilo considerare i profili di eventuali danni patrimoniali che potrebbero determinarsi a carico dei soggetti pubblici detentori di quote di partecipazione. In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 14.2 (testo 2 corretto), 15.18, 15.36, 18.8, 18.9, 15.87 (testo 3), 15.17 (testo 2), 15.0.500, 4.0.502, 5.501, 5.0.502, 5.0.502/100, 5.0.503, 8.0.500, 11.0.500, 14.0.500, 14.0.501,

15.500 (testo corretto) e 16.501 (testo 2); il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 19.7, 4.0.501, 15.3000/500 e 19.530. In ordine alla proposta 8.0.501, il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che dopo le parole: "n. 102," siano inserite le seguenti: "e nell'ambito del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto previsto dal predetto articolo 22, Il parere è di semplice contrarietà altresì sulle proposte 14.0.506, 14.0.507, 14.0.508, 14.0.509, 14.0.510,

15.526, 15.527, 15.528, 15.529, 15.530, 17.1 (testo 2), 18.502, 18.503, 18.504, 19.500, 19.501 e 19.502. Su tali emendamenti il parere di semplice contrarietà è reso con la segnalazione che l'approvazione di una di tali proposte determina l'assenza di copertura finanziaria delle restanti proposte recanti copertura rispettivamente a valere sulla tabella C, ovvero mediante aumento dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati. Il parere è sospeso sulla proposta 17.0.1/1, nonché su tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 19 e sui restanti emendamenti riferiti a partire dall'articolo 20 occorre che ci sia silenzio. Se volete che i lavori siano sospesi, stabilite voi, però così non ci sono le condizioni per andare avanti. Lo dico seriamente, perché non si riesce a seguire.

Onorevoli colleghi, prima di passare all'esame degli emendamenti presentati al decreto-legge in esame, do comunicazione all'Assemblea delle determinazioni assunte dalla Presidenza circa l'improponibilità di alcuni emendamenti. Il decreto-legge reca disposizioni per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, nonché altre disposizioni urgenti. Ai fini della valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti, anche alla luce delle decisioni prese dal Presidente della 1a Commissione permanente nel corso dell'esame in sede referente, la Presidenza si è attenuta ai seguenti criteri: conferma delle improponibilità già dichiarate in Commissione, salvo alcuni casi di significative riformulazioni dei testi; attinenza degli emendamenti al complesso delle materie trattate nel decreto; recepimento di ulteriori direttive urgenti;

in quanto già dichiarati improponibili in la Commissione: 4.0.500 del relatore, in materia di inquinamento acustico; 4.0.501 D'Alì, sulla nautica da diporto; in quanto introducono materie del tutto estranee al contenuto complessivo del decreto: 3.0.500 Pichetto Fratin, recante modifiche alla disciplina a favore di obbligazionisti e piccoli azionisti Alitalia; 4.0.502 D'Alia, in materia di fertilizzanti agricoli; 5.0.503 D'Alia, sulle società cooperative elettriche; 6.0.500 Zanoletti, che differisce 1'entrata in vigore di una norma già abrogata;

19.0.503 Fluttero, concernenti norme fiscali; 20.0.508 Barbolini, 20.0.505 Cutrufo e 20.0.506 D'Alia, sulla sicurezza operativa dell'ENAV; in quanto tendono a istituire nuove Autorità indipendenti o a sopprimere Autorità di ambito territoriale già esistenti: 5.501 Alicata; 15.91 Adamo, identico al 15.533 D'Alia. Infine, i seguenti emendamenti, già dichiarati improponibili in sede di 1a Commissione, sono stati ritenuti ammissibili in seguito all'introduzione nel testo dì espliciti riferimenti a procedure comunitarie: 5.500 (già 5.3) Fluttero, in materia di rifiuti apparecchiature luminose; 5.0.502 Governo (già 5.0.3 Zanetta), concernente ripristino risarcimento danno ambientale; 7.500 (già 7.10) Casoli, su promozione fonti rinnovabili; 19.0.501 (già 19.0.1) del relatore, su trasferimenti d'azienda e possibili ricadute sul personale;

è volto ad istituire l'Autorità di regolazione nell'ambito del servizio idrico. Sarebbe come se si dicesse che in presenza di una norma che liberalizza il settore del gas non è proponibile un emendamento che istituisce l'Autorità del gas.

è incompatibile con la presenza in questo decreto-legge di norme che liberalizzano il servizio idrico. Mi chiedo, signor Presidente, se non si debba riconsiderare questa decisione, tenuto conto nessuna iniziativa seria di liberalizzazione nel settore del servizio idrico potrà mai essere adottata se i soggetti interessati non avranno la garanzia, come accade per il settore del gas

sia un'Autorità terza rispetto ai soggetti che sono impegnati con interessi economici o sociali dati. Di conseguenza, ritengo che l'emendamento che istituisce l'Autorità sia perfettamente coerente con il contenuto di questo provvedimento. *(Applausi dal

chiedo, signor Presidente,

relativamente alle leggi di conversione di decreti-legge destinati ogni volta a rigonfiarsi impropriamente di norme non coerenti con il contenuto del decreto-legge stesso. Pur tuttavia, poiché abbiamo ritenuto in Commissione, dove pure è stato svolto un lavoro analogo da noi condiviso,

l'articolo 1 prevede che le imprese di autoriparazione debbano farsi carico di tutti gli oneri relativi allo smaltimento e alla gestione dei rifiuti dei veicoli

necessità di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia europea del 19 maggio 2009. La nostra proposta punta ad introdurre una maggiore severità sempre per porre all'attenzione il problema di eventuali conflitti di interesse. L'articolo 3, infatti, dispone l'esclusione dalla medesima gara di appalto delle imprese che si trovino legate da un rapporto di controllo,

che le imprese tra loro in rapporto di controllo possono essere ammesse a partecipare alla medesima gara di appalto a condizione che il rapporto di controllo non sia idoneo ad influire sulla formazione delle offerte o a determinare una turbativa di gara. Poiché

la possibilità della concorrenza, mentre nella formulazione adottata questa chiarezza si smarrisce.

l'articolo 3 regola le procedure di affidamento di opere pubbliche, servizi e forniture e prevede norme stringenti circa la partecipazione di ditte e di imprese alle gare. In particolare, impone che vi sia una netta indipendenza

È del tutto evidente la necessità di questo intervento atto a chiarire la norma e dare trasparenza ad un settore che, a torto o a ragione, è troppo chiacchierato. [DELLA

Il punto che critico è duplice. Da una parte, quello che tocca il comma 4 dell'articolo, là dove si prevede una deroga alla normativa ordinaria per un organismo che dovrà operare, tra l'altro, non in condizioni di urgenza e che è già stato inserito con grandi difficoltà in questa normativa che ci apprestiamo a trattare e successivamente ad approvare.

Ora si tratta, ad avviso mio e dei colleghi che hanno firmato l'emendamento, di una disposizione abbastanza vaga, anche perché nell'ambito degli appalti pubblici non abbiamo alcun punto di riferimento per stabilire quali siano le imprese

con un tempo quasi reale, un aggiornamento dei soggetti «con i quali non possono essere stipulati i contratti pubblici e successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetti lavori, servizi e forniture riguardanti le opere e gli interventi oggetto del presente articolo. In ogni caso, il mancato inserimento nella lista non esonera dal rispetto delle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252». Parliamo di un organismo che dovrà operare dal 2015. Non si vede l'urgenza di esonerarlo dal rispetto delle normative generali, a meno che non si voglia aggiungere qualcosa in più come controllo, che noi accettiamo e riteniamo utile ai fini antimafia. Soprattutto non capiamo con quale criterio potrebbe essere costituito l'elenco di imprese non soggette a rischio di inquinamento mafioso. Sarebbe invece molto più facile e soprattutto

quasi non conforme alla materia, mentre l'obiettivo perseguito si coniuga con quello, fondamentale, del rispetto dei principi comunitari e, in particolare, con quello richiamato dall'articolo 3, comma 1, lettera *g)*, della versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità economica Lo dico perché ho sentito nel corso del dibattito che tutti parlavano di un provvedimento sulle infrazioni comunitarie, mentre il provvedimento parla di «obblighi comunitari», che è cosa diversa. Gli obblighi

materia e della lotta alla criminalità organizzata. L'emendamento nasce proprio dall'utilità di fornire strumenti

non si vede perché non dovrebbe tentare di farlo anche a Milano in un'occasione di questo genere. Abbiamo utilizzato lo stesso modello usato per l'emergenza della ricostruzione dell'Abruzzo, dove già si era palesato questo rischio. Ad ogni modo, al di là di alcune valutazioni formali differenti, vorrei che l'Assemblea sapesse che questo emendamento in Commissione non ha registrato alcun voto contrario, avendo avuto i voti favorevoli della maggioranza e l'astensione dell'opposizione. Ne raccomando pertanto l'approvazione, data l'importanza che ha per un Paese come il nostro ospitare l'Expo 2015 a Milano.

3.0.7 (testo 2 )/1, perché la disposizione che lo stesso intende modificare prevede la creazione presso la prefettura di Milano di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso cui possano rivolgersi soggetti interessati. L'elenco è un'opportunità per le imprese esecutrici e le stazioni appaltanti in un'ottica di celerità e sicurezza delle procedure di individuazione dei contraenti. Tale strumento non è tuttavia la soluzione esclusiva, poiché le stazioni appaltanti possono, secondo i principi della libera concorrenza, individuare contraenti al di fuori di detto elenco, previa acquisizione delle necessarie informative antimafia. Il parere è contrario anche sul

L'ordine del giorno G3.0.101 della Commissione è stato approvato in Commissione e sottoscritto da tutti i Gruppi

nostro voto è favorevole nel merito. Esprimiamo, infatti, nel contempo la nostra critica più ferma, come da vari ambienti ormai viene testimoniato, per l'assenza e la mancanza di obiettivi prioritari

Con l'introduzione di questo subemendamento si potrebbe infatti garantire, senza soluzione di continuità, la possibilità di trasferire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le funzioni e i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore attribuiti all'ANAS ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e interamente partecipato dalle Regioni interessate o compartecipato dalle Regioni e dall'ANAS in misura non superiore al 50 A differenza della disciplina previgente, si prevede che la compartecipazione dell'ANAS a questo organismo di diritto pubblico non possa essere superiore al 50 per cento del capitale sociale. Questa disciplina potrebbe riuscire, da un lato, a garantire l'attuazione di un reale federalismo infrastrutturale - a cui i colleghi della Lega potrebbero essere interessati -volto anche a garantire una condizione specifica, cioè che le entrate legate ai pedaggi, per lo più provenienti dalla popolazione residente nel territorio, al netto degli investimenti e delle spese, rimangano sul territorio e, dall'altro, a contrastare il rafforzamento dei poteri dell'ANAS

la motivazione è analoga. Con l'introduzione degli emendamenti 3.0.5 (testo 2 corretto)/1 e 3.0.5 (testo 2 corretto)/3 si garantirebbe senza soluzione di continuità la possibilità di trasferire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le funzioni e i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore attribuiti all'ANAS ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e interamente partecipato dalle Regioni interessate o compartecipato dalle Regioni e dall'ANAS, eliminando il limite dell'esclusivo interesse regionale delle infrastrutture autostradali

gestione di infrastrutture autostradali. Le Regioni si sono attrezzate con l'ANAS, costituendo queste società ed iniziando a costruire e a gestire tratti di autostrada. Cosa accade a questo punto? Faccio un esempio che riguarda la mia Regione: penso alla penso alla tangenziale di Torino - ma potrei citare anche altre infrastrutture - che nel 2016 sarà un'opera ammortizzata, vale a dire un'opera che comunque ha smesso di costare e che comincia a rendere. Quello che si chiede con questo emendamento è proprio di assicurare,

onorevoli colleghi, il Gruppo del Partito Democratico voterà contro l'emendamento 3.0.5, anche nella sua versione corretta, non senza segnalare quattro aspetti all'attenzione della Presidenza e dell'Assemblea. La prima questione è già stata adeguatamente esposta, e non solo per questo dispositivo, dal senatore Ceccanti in occasione dell'illustrazione della pregiudiziale, per un evidente vizio di costituzionalità nell'uso assolutamente improprio dell'articolo 77 della già evidenziato nel titolo stesso dell'emendamento, laddove si parla di adeguamento alla disciplina comunitaria e non di correzione della stessa; di fatto, un'interpretazione facoltativa, non imposta, né richiesta dalla comunità, circostanza che poteva giustificare la necessità e l'urgenza del provvedimento in questione. Una seconda questione che voglio ulteriormente evidenziare è quella dell'ammissibilità dell'emendamento presentato. Un emendamento non urgente e non necessario, che ha espropriato la competenza specifica dell'8a Commissione, che di fatto ha assistito, come purtroppo altre volte, da spettatore passivo (analogamente a quanto già successo recentemente per il trasporto universale ferroviario), nonostante lo specifico lavoro da essa svolto; ciò avrebbe probabilmente richiesto una censura di merito e di metodo da parte della Presidenza. Una terza questione, che è quella centrale nell'emendamento in questione, è nel tentativo, come è stato ricordato, di esproprio postumo da parte dello Stato ai danni delle Regioni sul federalismo infrastrutturale, già avviato in alcune delle nostre Regioni proprio per effetto del provvedimento presente nella finanziaria 2008. Ciò, peraltro, era tanto più ravvisabile nell'originaria stesura dell'emendamento, che tradiva le sue reali intenzioni traducendo in maniera più rozza i concreti orientamenti di un Governo proteso con ogni mezzo a fare cassa, in palese contraddizione con lo spirito federalista, che propugna a parole ma che nega, come può, nei fatti e negli atti, con buona pace dei colleghi leghisti. In ultimo, come ha dimostrato palesemente anche il precedente ordine del giorno accolto dalla Commissione, l'emendamento così formulato non tiene conto delle specificità territoriali, che non sempre vedono coincidere le infrastrutture con gli ambiti esclusivi di una sola Regione, come nel caso della autostrada A4, del tronco Venezia-Trieste, che evidentemente insiste su due Regioni e non su una.

**Il Senato non approva.**

senatori Segretari, a votare per se stessi. Sono scene che non cambiano i risultati e danneggiano il prestigio del Senato.

tra di noi c'è stato francamente un certo stupore perché il collegamento della norma - che poi la Commissione ha votato - con il decreto-legge è, collega Vizzini, coraggioso

In queste ultime settimane autorevoli magistrati che ogni giorno combattono con coraggio la criminalità mafiosa hanno evidenziato il rischio di una pesante infiltrazione della criminalità organizzata, non solo della mafia e di Cosa nostra, ma della camorra, della 'ndrangheta e di altre organizzazioni criminali, anche di nuovo conio, nei confronti degli appalti pubblici, soprattutto nel settore delle grandi opere.

di infrastrutture necessarie per ospitare l'Expo di Milano fra qualche anno. Si tratta di un tema serio, ed è la ragione per la quale

Se è vero che c'è un allarme così forte, colleghi, la strada maestra per affrontarlo non è quella di norme speciali che di volta in volta vengono approvate. Di specialità il nostro Paese non ne può più.

Tuttavia, il metodo della specialità sta diventando lo strumento con cui si aggirano gli ostacoli e si pensa di risolvere i problemi.

Presidente, sappiamo perfettamente che a Milano già ci si sta muovendo, indipendentemente dalla legge, per attrezzarsi a contrastare questo rischio; sappiamo che la DIA segnala ordinariamente alla procura e alla prefettura i rischi di possibili imprese mafiose che operano in questo campo; sappiamo che la procura stessa si è attrezzata per contrastare problemi di questo tipo. I senatori del Partito Democratico, in considerazione della delicatezza dell'argomento, non voteranno contro

ordinaria per contrastare un fenomeno che non riguarda solo l'Expo di Milano, ma tutte le grandi opere del Paese. Scorciatoie, Presidente, non esistono. Ecco la ragione per la quale, pur manifestando attenzione con l'astensione, i colleghi del Partito Democratico non possono votare a favore dell'emendamento in

il decreto ministeriale sull'ambientalizzazione deve essere ricondotto ad un impianto razionale più compatibile con l'ordinamento. Che senso ha prevedere un *iter* accelerato per l'adempimento di obblighi già previsti dalla legge vigente? è necessario che le linee guida stabiliscano standard più elevati di quelli attualmente previsti - come stabilisce l'emendamento 4.11 - ai fini dell'attribuzione di un beneficio agli impianti. Inoltre,

di coefficienti e parametri ambientali - che, per la verità, non sono meglio precisati - cui riconnettere il dimezzamento dei tempi per l'autorizzazione, oltre a prevedere il concerto con il Ministero dello sviluppo

il decreto ministeriale di cui all'articolo 4 nella sua fase applicativa è suscettibile di incidere su una materia che è stata oggetto di legislazione primaria, riguardante anche i tempi di realizzazione degli impianti. l'emendamento introduce una clausola di salvaguardia che preveda il parere delle competenti Commissioni parlamentari. L'emendamento 4.14 L'emendamento 4.14 punta ad ancorare i benefici ai soli impianti che siano in regola con le leggi nazionali e comunitarie, al fine di evitare che la scelta di alcuni parametri e coefficienti in sede di decreto ministeriale possano privilegiare impianti non ottimali. L'emendamento prevede inoltre il rispetto della legislazione regionale e il riconoscimento della competenza sancita dal Titolo V della Costituzione. L'emendamento 4.15 con semplicità esclude il dimezzamento dei tempi previsti dal comma 4 per gli impianti nucleari a causa della loro complessità. L'emendamento 4.16 propone di recuperare, in termini di maggiore responsabilizzazione, un ruolo delle Regioni (quindi è collegato all'emendamento precedente) e degli enti locali in materie anche di loro competenza, come la localizzazione degli impianti, le osservazioni tecniche relative all'impatto sull'ambiente e sulla salute dei cittadini, al fine di evitare che i tempi dimezzati non consentano loro di esprimersi in materia. L'emendamento 4.17 è volto a prevedere con maggiore chiarezza una competenza regionale e degli enti locali con riferimento al comma 5, riguardante la Conferenza dei servizi. L'emendamento 4.19 esclude la ricorribilità ai commissariamenti speditivi previsti dalla legge 3 n. 102, per gli impianti nucleari, in ragione della loro complessità e della loro peculiarità nell'impatto sull'ambiente e sulla sicurezza dei cittadini.

4.25, che ha contenuti analoghi all'emendamento 4.15 di cui è primo firmatario il senatore Pardi, sostanzialmente si chiede di escludere dalle semplificazioni delle istruttorie sulla compatibilità ambientale degli impianti delle infrastrutture energetiche quelli per la produzione di energia nucleare. Faccio presente che questa richiesta è stata condivisa all'unanimità dalla Commissione ambiente, come può

Pardi. Ne devo dedurre che il Governo è intenzionato a utilizzare procedure semplificate per quanto riguarda in particolare le autorizzazioni ambientali nel momento in cui dovesse decidere di realizzare centrali nucleari. Ne prendiamo atto.

condizionato da parte della Commissione bilancio, la quale ha chiesto di aggiungere, dopo le parole «n. 102», le parole: «e nell'ambito del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto previsto dal predetto articolo 22,

il parere è favorevole.

Questa parte prevede la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica col fine di promuovere lo sviluppo economico, civile e sociale delle collettività territoriali. principi ai quali si ispira la materia sono la tutela della concorrenza, la libertà di stabilimento, la libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale di rilevanza economica in ambito locale, nonché la garanzia del diritto di tutti gli utenti all'universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere *e)* ed *m)*, della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, proporzionalità e leale collaborazione.

riconosciuto il relatore, assolutamente risolto e che non crediamo possa essere risolto con un articolo inserito un po' di soppiatto rispetto ad una materia così importante, nientemeno che in un decreto e nemmeno in una legge comunitaria. Il problema dei servizi pubblici locali è di grande rilevanza, anche in rapporto alle tematiche che dovranno essere affrontate a seguito dei decreti attuativi sul federalismo fiscale. sembra veramente un fatto poco corretto anche nei riguardi del Parlamento inserire un articolo del genere in un decreto che non offre nemmeno la possibilità di riflettere su tematiche di così grande interesse, di carattere sociale e anche di rilievo economico.

ho parlato con il presidente Schifani della questione che lei aveva sollevato in merito all'emendamento 15.91 della senatrice Adamo. pertanto le determinazioni del Presidente. La Presidenza non può che ribadire sul piano formale che sulle questioni di di proponibilità e ammissibilità la Presidenza stessa decide, sulla base dell'articolo 97 del Regolamento, in modo inappellabile. Questo dunque da un punto di vista formale di procedura. Da un punto di vista sostanziale, la Presidenza conferma la giurisprudenza costante di questa legislatura, secondo cui ai decreti-legge non sono proponibili emendamenti di carattere ordinamentale come quello in questione. La Presidenza ritiene che un tale orientamento, fatto valere in passato anche nei confronti di emendamenti del Governo e della Commissione, sia in primo luogo una garanzia del Senato stesso verso un

Signor Presidente, vorrei citare le parole dello studente iraniano Mahmoud Vahidnia: «Io non ho mai visto nessuno criticarla pubblicamente. Perché nessuno può permettersi di criticarla in questo Paese?». Lo scorso 28 ottobre

gradualmente si tinge di cattive intenzioni». Questa critica pacata nei toni, ma serrata, ha suscitato qualche giorno fa tra i presenti applausi prima timidi e poi entusiasti, perché egli

Il mondo libero non può non preoccuparsi dei giovani iraniani assetati di democrazia, di modernità, di libertà, come hanno dimostrato i disordini dello scorso giugno, soffocati, come tutti sappiamo, nel sangue.

uno dei più importanti centri di ricerca europei, il più importante italiano, azienda che purtroppo non naviga in buone acque. Vorremmo sapere dal Governo